Comunico che in data 11 aprile 2011 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze:* «Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011» Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 20 aprile. Restano confermati gli argomenti già previsti dal calendario della settimana corrente. Il calendario della prossima settimana prevede l'esame del decreto-legge recante interventi in favore della cultura e altre disposizioni urgenti,

per l'elezione dì un giudice della Corte costituzionale. La chiama comincerà dagli onorevoli senatori. La seduta dell'Aula avrà inizio pertanto alle ore 10. Nella settimana tra il 25 aprile e il 1° maggio 1'Assemblea non terrà seduta. Le Commissioni potranno convocarsi in relazione alle esigenze dei rispettivi programmi dei lavori. La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre convenuto che il Documento di economia e finanza - previsto dalla legge di riforma di contabilità e finanza pubblica - sarà inserito nel calendario dei lavori non appena trasmesso dal Governo e nel rispetto dei tempi

del Governo, onorevoli senatori, la 13a Commissione permanente ha elaborato in sede referente il testo in esame confermando le principali scelte normative proposte dal Governo e apportando al contempo ad esse tutte quelle modifiche ed integrazioni che sono risultate opportune al termine di un confronto attento e approfondito, che ha visto i Gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, fornire il loro attivo contributo ai lavori, anche attraverso rilevanti proposte emendative, e concordare sui contenuti del testo da sottoporre all'Assemblea.

di cui all'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, che viene di conseguenza abrogato. Le nuove disposizioni in tema di «Giornata nazionale degli alberi» appaiono necessarie per superare talune criticità normative registratesi nell'esperienza attuativa della precedente festa, soprattutto a causa dell'estrema genericità della norma istitutiva, che risale al lontano 1923, e del suo carattere di mero stimolo di iniziative volontarie degli istituti scolastici, peraltro con copertura finanziaria imprecisata. Il superamento delle criticità normative esistenti può consentire il rilancio di un momento simbolico e celebrativo di antica tradizione - l'«*Arbor Day*» venne celebrato per la prima volta in Nebraska (USA) il 10 aprile 1872 e in Italia la «Festa degli alberi» è stata istituita alla fine dell'Ottocento da Guido Baccelli e tenuta per la prima volta nel 1898 - che mantiene tuttora l'intera sua vitalità ed anche una rinnovata attualità. Difatti, la «Giornata nazionale degli alberi» si inserisce oggi nel più ampio quadro delle azioni intraprese al fine di diffondere tra le nuove generazioni la consapevolezza dell'assoluta necessità di salvaguardare e valorizzare l'ambiente e il patrimonio arboreo e boschivo, di ridurre le emissioni inquinanti, di prevenire il dissesto idrogeologico e di migliorare la qualità dell'aria. Inoltre, con l'articolo 2 del disegno di legge si modificano alcune disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, che ha introdotto l'obbligo in capo ai Comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente. Si tratta di modificazioni finalizzate a conferire maggiore effettività all'obbligo di messa a dimora sia riducendo i relativi termini da un anno a tre mesi, sia creando i presupposti affinché gli amministrati possano conoscere se e in che misura, in ciascuna consiliatura, quest'obbligo sia stato rispettato dagli amministratori di ciascun Comune, attraverso l'introduzione del bilancio arboricolo. La Commissione ha approvato alcune proposte emendative dirette a modificare l'articolo 2 del testo presentato dal Governo in alcuni specifici punti, allo scopo di precisare che l'obbligo di messa a dimora sussiste solamente per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e che il termine di tre mesi si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione, fermo restando che la messa a dimora può comunque essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. La Commissione ha altresì modificato la disciplina relativa al bilancio arboricolo del Comune, nel senso di prevedere che tale documento deve anche dare conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di competenza comunale. La Commissione, in osservanza del parere reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5a Commissione permanente, ha poi approvato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 3 del disegno di legge. che rivestiva comunque una collocazione marginale rispetto all'oggetto e alle finalità del provvedimento, prevedeva l'esenzione dalla TOSAP, di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo n. 507 del 1993, per le aiuole realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi allo scopo di incentivare la trasformazione in aiuole articolo 3 nel testo della Commissione) modifica l'articolo 43 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, inserendo alcuni nuovi periodi dopo il primo periodo del comma 2 del medesimo articolo 43. L'articolo 43 della citata legge n. 449 prevede, al comma 1, che, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Il primo periodo del comma 2 del medesimo articolo specifica che le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. 3 del Testo della Commissione del disegno di legge in esame si stabilisce che rientrano nell'ambito di tali iniziative anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica Il testo originario del provvedimento faceva riferimento al patrimonio arboreo della città, ma la Commissione ha approvato una proposta emendativa che, più propriamente, fa invece riferimento al patrimonio arboreo delle aree urbane. Sempre attraverso la modifica recata dall'articolo 3 del Testo nel caso di iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica, il Comune possa inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti devono essere definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza unificata, entro giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame. La Commissione ha approvato tre emendamenti volti a introdurre tre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 del disegno di legge nel Testo della disposizioni per la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, e stabilisce che le Regioni, le Province e i Comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, adottano misure volte a favorire l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento: alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio, il drenaggio delle acque piovane e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia; agli edifici esistenti, tramite la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici; alle coperture a verde di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili; al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale. Commissione detta disposizioni in materia di incentivi all'utilizzo del verde pensile e al comma 1 prevede che le amministratori comunali, con appositi regolamenti, adottino le necessarie disposizioni riguardanti gli edifici di nuova costruzione allo scopo di favorire l'utilizzo di tecniche che prevedono il ricorso al verde pensile e alle pareti rinverdite. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che le recinzioni di stabilimenti industriali o commerciali di nuova edificazione devono prevedere il ricorso a soluzioni che utilizzino il verde pensile e le pareti rinverdite. Il comma 3 introduce una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 45.000 euro, da ripartire in in dieci quote annuali di pari importo, per le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2011, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti, unità immobiliari o recinzioni, riguardanti tetti, coperture o pareti esterne e rappresentate dalla realizzazione del verde pensile e delle pareti rinverdite. Il comma 4 affida ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di fruizione degli incentivi previsti dal comma 3. Il comma 5, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri, che ci riserviamo di valutare in

alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale. Al comma 1, esso stabilisce la definizione di «albero monumentale» e, al comma 2, affida ad un decreto interministeriale, emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento ad il periodico aggiornamento degli elenchi regionali e comunali. Le Regioni, ai sensi del comma 3, recepiscono la definizione di albero monumentale recata dall'articolo 6, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai Comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. Il comma 4, infine, prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali. Sono fatti salvi, però, gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. e media - 7 Istituto comprensivo «Giuseppe Aurelio Costanzo» di Siracusa, ai quali do il benvenuto

Presidente, sono lieto di questa iniziativa del Governo, che, attraverso il lavoro che è stato fatto, come riassunto dal collega

di tanti nostri concittadini e alle tradizioni proprie di tutti i nostri territori. Sono anche lieto che questo provvedimento aggiorni una legge che porta la mia firma, approvata nel lontano 1992, che sta per compiere vent'anni e che ha conosciuto un'applicazione discontinua: una legge che nasce da una intuizione, condivisa da tante associazioni ambientaliste e amministrazioni locali, e che ha un significato simbolico, prevedendo la messa a dimora di un albero

fortuna e attenzione, legata anche ad un modesto finanziamento annuo disponibile, poi ripartito dalla Conferenza Stato-Regioni

Complessivamente, si deve riconoscere l'importanza della nostra potente, formidabile struttura arborea della forestazione e in generale dell'evoluzione delle aree verdi urbane e periurbane come uno degli aspetti più importanti, signora Presidente, della qualità della vita e del rapporto della nostra società con la natura. Anche da questo punto di vista è molto significativo che al centro di questa normativa vi sia l'aggiornamento di una cerimonia tradizionale varata dal fascismo, che oggi con il provvedimento che ci accingiamo ad approvare, conosce non solo un aggiornamento ma anche un ripensamento significativo. È chiaro che l'importanza del patrimonio arboreo e boschivo vale per i fini paesaggistici, ambientali e di igiene urbana, ma aggiungo che mi piacerebbe venisse recepita all'articolo 1, collega Leoni, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana. Le culture dei nostri territori conoscono una simbologia legata agli alberi, alle piante e alle coltivazioni che è eterna.

che sono da tutelare esattamente come dei monumenti, con la differenza che sono dei monumenti viventi, e dunque qualcosa che si lega in molti casi a tradizioni, simbologie e realtà storico-culturali proprie dei nostri territori. Tutti convengono sui benefici degli alberi per la qualità dell'aria, per ridurre l'inquinamento e rendere più vivibili gli insediamenti urbani, sono determinanti in una corretta organizzazione dell'assetto idrogeologico del territorio, e infine concorrono in modo significativo con le politiche di forestazione ad assorbire la CO2, e dunque concorrono a loro volta al conseguimento degli obiettivi che anche il nostro Paese ha assunto per quanto riguarda la riduzione delle emissioni clima-alteranti, in particolare, quelle riferibili al Protocollo di Kyoto e agli accordi internazionali sul clima. «Non è l'Italia» - diceva Varrone nel «*De re rustica*» - «piantata ad alberi in modo da sembrar tutta un frutteto?». Oggi l'Italia non è ovviamente più questa, o solo questa; tuttavia, il senso e il valore degli alberi e la divulgazione della loro funzione, il senso della relazione tra gli alberi e la persona ha spesso assunto un valore spirituale, spirituale, ma anche un valore come quello che - e concludo - un grande scrittore quale Ennio Flaiano, nel «Diario notturno», così descriveva: «La saggezza di certi vecchi alberi mi riempie di venerazione. Ognuno, credo, è legato agli alberi della sua terra, come ogni uomo si accorge, un bel giorno, di essere suo padre e suo nonno e che questa è l'unica e che questa è l'unica immortalità possibile». Non so se sia l'unica immortalità possibile; certamente è il senso di una continuità della vita dell'uomo sulla terra, del suo rapporto con la natura che con questa normativa può senz'altro

Presidente, gentili colleghe e colleghi, istituire, come si intende fare con questo disegno di legge, la «Giornata nazionale degli alberi» è opera assolutamente meritoria, per diversi motivi. Nel nostro Paese, nonostante l'impegno e gli sforzi di associazioni - prima tra tutte Legambiente - che lavorano da anni per questo obiettivo, le potenzialità della risorsa ambiente non sono ancora valorizzate *in toto*, e lo sviluppo cosiddetto sostenibile è un terreno poco praticato.

Anche nella prospettiva del pacchetto clima «20-20-20», credo che questo disegno di legge vada in quella direzione. E allora, un provvedimento normativo come quello al nostro esame, finalizzato a creare maggiori spazi verdi nelle aree urbane, può rappresentare un passo importante sulla strada del radicamento di una cultura ambientale più responsabile e matura. Diffondere tra le giovani generazioni la consapevolezza della necessità improcrastinabile di salvaguardare e valorizzare il patrimonio arboreo e boschivo, di ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare la qualità dell'aria è fondamentale; per non parlare dell'importanza di potenziare il patrimonio boschivo per prevenire il dissesto idrogeologico, vista la natura del nostro Paese. Il rischio idrogeologico interessa una parte considerevole del territorio nazionale e, vale la pena ricordarlo, è fortemente condizionato anche dall'azione dell'uomo e aggravato dal continuo disboscamento.

Credo che anche dal disegno di legge oggi in discussione possa venire un contributo importante per cominciare ad intervenire con un'azione complessiva su questo versante per mettere in sicurezza il territorio nazionale. Ma valorizzare l'ambiente è anche opera culturale. In questo senso, acquisisce importanza ancora più rilevante la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale e storico, al centro dell'emendamento da me presentato e recepito dal relatore - cosa che noi apprezziamo moltissimo - anche al fine di recuperare memoria e storia attraverso gli alberi. Penso ai cosiddetti giganti, gli alberi ultrasecolari presenti nel Parco nazionale della Sila - e in tanti altri nel nostro Paese - e al fatto che una ricchezza così importante, anche ai fini dello sviluppo turistico, sia molto poco nota, e noi dobbiamo incentivare anche questa cultura. L'archivio realizzato dall'associazione «Patriarchi della natura in Italia», alla data del 20 luglio 2010 conta 8.245 elementi e comprende tutte le piante delle quali si è avuta segnalazione dal 1980 ad oggi. Negli ultimi 30 anni alcune sono purtroppo già morte o versano in pessime condizioni (al momento sono 153). Pertanto, le piante ancora in vita o delle quali, successivamente

pertanto un'azione complessiva, basata su rilevamenti ed analisi dell'esistente ed è chiaro che, da solo, il disegno di legge che istituisce la «Giornata degli alberi» il 21 novembre non segnerà un punto di svolta. come ho già detto, se accolto da Regioni e Comuni, dalla società e dalla sensibilità di tante associazioni culturali, con lo spirito che ha animato il legislatore nel redigerlo, esso può rappresentare un primo passo per far maturare una nuova consapevolezza,

il *modus operandi* imposto in questi mesi alla nostra Assemblea dal Governo e dalla sua maggioranza consente l'approdo in Aula di ben pochi disegni di legge di iniziativa parlamentare e - in aggiunta - il positivo esito ne è garantito solo se largamente condivisi. Questo è il caso odierno, che sconta peraltro un'altra evenienza tipica delle circostanze operative attuali, vale a dire quella di dover caricare un testo di ogni possibile argomento per poter portare all'attenzione dell'Assemblea temi rilevanti, non diversamente segnalabili. Del resto, se non fosse per la soddisfazione derivante dal vedere trattato oggi in Aula questo disegno di legge, elaborato nella Commissione della quale sono componente, mi sentirei di chiedere ragione dell'inspiegabile rallentamento del ritmo dei nostri lavori d'Aula, così confliggente con quello, invero incalzante in questi ultimi giorni, dell'Aula della Camera dei deputati, dovuto forse all'interesse diretto del signor Presidente del Consiglio per i temi colà trattati, su istanza del suo Governo. basta volerlo: si può dare consistenza ad un ordine del giorno per l'Aula, e credo sarebbe elegante per la maggioranza dare dimostrazione di positiva volontà di legiferare anche su temi non di stretta utilità e pertinenza del suo principale referente. Ci sono molti disegni di legge predisposti, ma dormienti fra il livello delle Commissioni e quello dell'Aula. Da senatore semplice, avrei piacere che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi si occupasse approfonditamente della questione, forzando resistenze esterne e riappropriandosi della facoltà di rendere più intensi i nostri lavori d'Aula. Non è quindi negativo che il disegno di legge in esame, di cui è relatore il collega Leoni, originariamente volto a disciplinare in modo aggiornato - da un lato - la ben nota Festa degli alberi e -

circostanze specifiche, sia stato arricchito in Commissione da alcuni emendamenti aggiuntivi, che hanno ampliato la portata del medesimo su un tema di assoluto significato socio-ambientale. Mi promozione degli spazi verdi urbani, all'incentivazione per l'utilizzo del verde pensile e alla definizione degli alberi secolari e monumentali da tutelare. Nel complesso, si tratta quasi di un breve testo unico, che riassume orientamenti ed indirizzi altamente positivi per l'ampliamento e la valorizzazione del verde nei contesti ove abitiamo, sia con intervento diretto degli enti pubblici competenti, sia prevedendo le diverse forme di attivo coinvolgimento del privato.

alla natura che è contenuto in questo disegno di legge è ispirato anche dal fatto che c'è un rapporto simbolico tra politica e natura: edera, margherita, quercia, ulivo, garofano, e buon'ultima anche la rosa nel pugno sono stati simboli della politica,

Sicuramente, quindi, occorre mantenere l'attenzione al rapporto con l'ambiente e cercare quanto più possibile di collegare l'aspetto simbolico che ha questo disegno di legge con una serie di ulteriori di ulteriori misure, che abbiamo cercato di elaborare anche con degli emendamenti che illustrerò più avanti, che devono tenere in considerazione il fatto che la sola aggiunta di un albero ogni qualvolta nascano una bambina o un bambino non va nella direzione dello sviluppo degli spazi verdi urbani. che deve essere perseguito con grande urgenza e altrettanta necessità, occorra adottare delle norme relative alla cosiddetta rottamazione edilizia:

una serie di misure che devono essere promosse verso l'ipotesi della cosiddetta rottamazione edilizia, sulla quale il Governo ha espresso un parere favorevole.

fatto di vere e proprie megalopoli: se si prende l'automobile e si va da Roma a Salerno, si noterà che non esiste soluzione di continuità tra costruzioni, e quindi occorre recuperare le aree le aree protette, i parchi urbani o, per così dire, extraurbani, che in virtù dell'esistenza delle megalopoli non esistono più. Nell'ordine del giorno chiediamo anche di presentare una riforma della legge quadro sulle aree protette che ridefinisca il sistema delle entrate da destinare al conseguimento dei fini istitutivi dei parchi e delle riserve statali e regionali, assoggettando la realizzazione delle operazioni di trasformazione urbanistica ed edilizia trasformazione urbanistica ed edilizia eseguite all'interno di ambiti territoriali che nel loro complesso traggono vantaggi e benefici di diversa natura dalla presenza delle aree protette a una forma di prelievo speciale, e vincolando il gettito di quest'ultimo al finanziamento di un processo di acquisizione delle aree comprese nei parchi e nelle riserve naturali al patrimonio degli stessi enti di gestione, ovvero alla creazione di un soggetto istituito *ad hoc* con questo mandato esclusivo, sul modello di alcuni enti già esistenti in Italia, come ad esempio quello relativo alla conservazione delle coste della Sardegna, o come quelli che esistono già da più di trent'anni in Francia; a promuovere, attraverso le opportune intese con le Regioni, una revisione del sistema degli oneri cui sono soggetti quanti realizzano trasformazioni del territorio che riducono la dotazione di aree libere ovvero non urbanizzate dei Comuni, introducendo a carico dei soggetti richiedenti il titolo abilitativo l'obbligo di realizzare controprestazioni ecologiche, appropriate alle diverse

al finanziamento di programmi regionali e comunali locali per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle aree non urbanizzate, per la pianificazione e la gestione durevole di ambiti di riserva, di corridoi e discontinuità ecologiche, di cui

che si aggancia ad un simbolo, per quegli impegni che il Governo, non necessariamente attento a questa fase del dibattito, dovrebbe assumersi per la tutela del territorio. Quindi, riteniamo necessario impegnare i Comuni e le Province all'obbligo di adottare sistemi di contabilità ambientale ed urbanistica, attraverso i quali dare conto delle prestazioni che questi livelli di governo ogni anno assicurano in fatto di contenimento ovvero di riduzione delle aree urbanizzate, di gestione e messa in sicurezza delle aree libere (aree agricole, zone comprese in parchi e/o riserve, ambiti a diverso titolo non urbanizzati e non urbanizzabili) e di acquisizione e sistemazione delle aree destinate dalla strumentazione urbanistica vigente a verde pubblico. Si tratta, forse, di ampliare lo spettro degli impegni da assumersi in questa situazione, ma proprio perché, come diceva il senatore Rutelli, primo intervenuto in questa discussione generale, qui si parla anche di qualità della vita, la cementificazione è il peggiore nemico che possa esserci nella qualità della vita. Piantare un albero ogni qualvolta nasce una bambina o un bambino, specie in un momento storico italiano dove c'è un decremento delle nascite, potrebbe non essere neanche più simbolicamente sufficiente. Occorre, quindi, assumersi degli impegni un po' più

onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, l'Italia dei Valori condivide la finalità di perseguire, attraverso il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo,

Pertanto, come ampiamente documentato dalle mozioni che abbiamo presentato in materia di politiche di riduzione delle emissioni di gas serra, condividiamo ogni iniziativa volta sensibilizzare e coinvolgere i cittadini e le amministrazioni riguardo al problema della CO2 e al contributo che le aree verdi urbane possono offrire in tal senso, specialmente nelle aree urbane. Queste, infatti, per la maggior densità abitativa e concentrazione di attività, sono soggette al fenomeno della cosiddetta isola di calore, che determina, insieme all'inquinamento, temperature sensibilmente più alte che nelle aree periferiche e periurbane.

anche le iniziative sulla sensibilizzazione ed educazione alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al miglioramento della qualità dell'aria: dobbiamo, però, registrare che una nostra mozione di indirizzo in materia, come anche gli emendamenti da noi presentati in sessione di bilancio, sono restati lettera morta. Vorremmo, in altre parole, che attività più fattive prendessero il posto delle mere celebrazioni, come quella che, pur lodevolmente, si vuole qui istituire all'articolo 1. Con l'occasione, mi sembra doveroso segnalare un emendamento al comma, 1 che non ne altera il contenuto ma lo riscrive in forma più logica dal punto di vista delle regole legislative. Il dibattito in Commissione ha visto accolte molte proposte migliorative delle opposizioni, volte da un lato a rendere fattibile la disciplina sulla messa a dimora dei nuovi alberi già prevista oggi dalla legge (evitando, ad esempio, di spendere denaro per piantare alberi fuori stagione che poi sarebbero inevitabilmente morti) e, dall'altro, ad arricchire il contenuto del disegno di legge in materia di tutela delle alberature monumentali e di verde pensile. In materia di sponsorizzazioni riteniamo utile l'integrazione proposta all'articolo 43 della legge finanziaria per il 1998, purché sia chiaro (abbiamo sia un emendamento che un ordine del giorno in tal senso) che le iniziative sulla CO2 debbono rispettare gli stessi requisiti delle altre: vale a dire, essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e comportare risparmi di spesa per le pubbliche amministrazioni. Poiché la formulazione testuale dell'articolo 3 lascerebbe ipotizzare una dichiarazione *ope legis* di assolvimento di tali requisiti, abbiamo presentato un emendamento chiarificatore ed un ordine del giorno, qualora non si volesse modificare il testo uscito dalla Commissione. Allo stesso modo ci pare saggio chiarire che le iniziative di sponsorizzazione non attribuiscono alcun titolo all'utilizzo esclusivo di un bene pubblico a fini pubblicitari o commerciali e che restano fermi, ove presenti, i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela sulle aree verdi previste dalla normativa vigente. Con riferimento all'articolo 4, sulle iniziative locali, ci sembra opportuno che già nel comma 1 si specifichi la finalità di perseguire il risparmio e l'efficienza energetica, visto che la lettera *c)* successivamente ne fa cenno. Sull'articolo 5, riguardante il verde pensile, abbiamo invece una perplessità: il secondo comma, per come è scritto, afferma che le aziende «devono prevedere il ricorso a soluzioni» di tal genere per i nuovi stabilimenti. Poiché si pone un obbligo, cui corrisponde un beneficio fiscale con oneri cui si fa carico attraverso il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, vi è il rischio che questa categoria di beneficiari assorba l'intero ammontare dei 10 milioni messi a disposizione dalla legge. In ogni caso, sempre al fine precauzionale di evitare localmente utilizzi impropri di soluzioni di per sé assolutamente benefiche, ci sembra opportuno, al primo comma, suggerire l'opportunità di ribadire espressamente la normativa vincolistica o di tutela eventualmente presente sul bene o sull'area in cui il bene ricade. In ogni caso, si può dire sin da ora che, condividendo le misure proposte dal disegno di legge e tenuto conto del fatto che gli emendamenti sono animati da uno spirito di ragionevolezza e attenzione alle ricadute concrete della norma una volta licenziata definitivamente, annunciamo - e mi rivolgo al relatore - che ove il loro inserimento nel testo fosse ritenuto tecnicamente non fattibile in questa fase, si può procedere alla loro trasformazione in ordini del giorno.

esaminato il presente disegno di legge, ha già approvato un nostro ordine del giorno in cui, tenuto conto del fatto che il Fondo istituito dalla finanziaria 2008 per il verde urbano non risulta essere stato rifinanziato, si impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative per il finanziamento delle attività di incremento del patrimonio arboreo, finalizzate a migliorare la qualità dell'aria e del paesaggio e a ridurre le emissioni di CO2, mediante la realizzazione e la cura di nuove aree verdi in zone urbane, con particolare riferimento ai Comuni a maggiore crisi ambientale e a quelli a maggior indice di densità abitativa o di edificazione dei suoli. poiché attualmente nelle nostre città molti giardini, ville e parchi versano in una situazione di difficoltà - se non di degrado - ed è invece necessario assicurare il decoro e l'ottimale gestione di giardini che, oltre oltre ad offrire un positivo impatto ambientale, rappresentano di per sé una meta di attrazione turistica, chiediamo al Governo, sensibilizzando i Comuni, di assicurare manutenzione, conservazione e restauro, fruizione pubblica e riqualificazione degli spazi verdi esistenti nelle città, con particolare attenzione per i parchi e i giardini storici. In tale contesto, particolare attenzione andrebbe rivolta alle operazioni di potatura, che vanno effettuate periodicamente, e che spesso lasciano molto a desiderare per il modo sbrigativo in cui le si realizza, anche fuori stagione. È infatti importante che le varie misure di incentivo per la piantumazione di nuove alberature non facciano da disincentivo alla tutela di quelle esistenti o alla sostituzione delle alberature abbattute o malate, che comunque debbono essere assolti nella ordinaria amministrazione. Ci auguriamo che il presente disegno di legge costituisca l'occasione comunque per pensare ad un rilancio della bioedilizia e della bioarchitettura, affinché anche nella pianificazione urbana si preveda obbligatoriamente la progettazione e la realizzazione di nuovi ampi spazi di verde pubblico. Così facendo, anche le città del domani potranno usufruire di quei grandi polmoni verdi e di quei parchi di cui oggi fortunatamente disponiamo, almeno per le parti che si sono salvate dall'urbanizzazione di fine Ottocento e del Novecento.

infatti, il comportamento di tutti quei bambini che sono diventati adulti e che dovevano occuparsi di alberi e di ambiente nel nostro Paese, gli esiti sono stati talvolta incerti, quando non completamente negativi.

che prevede una serie di disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale,

oggi, per ripiantumare il gelso - un albero che appartiene alla tradizione culturale lombarda, perché era l'elemento fondamentale per la produzione della seta

accanto a chi amministra, accanto a chi, come noi, fa politica, accanto a tutti coloro che di verde, di vivibilità e sostenibilità ambientale devono occuparsi. come è stato correttamente ricordato dal relatore, il disegno di legge oggi all'esame del Senato interviene su una normativa già esistente,

imponendo e prescrivendo un controllo e un obbligo di comunicazione rispetto agli adempimenti che in essa sono individuati, cioè l'adempimento di piantare un'essenza legnosa, un albero, in occasione della nascita di ogni bambino.

la necessità che le piantumazioni avvengano secondo il ciclo naturale delle piante (introducendo quindi un contenuto ambientale) che i Comuni di piccole dimensioni possano essere esonerati da un obbligo prescrittivo, non già perché ad essi non compete la tutela dell'ambiente urbano e delle emergenze positive dal punto di vista ambientale e naturalistico, ma perché nei territori dei piccoli Comuni va garantita e valorizzata la fruizione dello spazio verde e naturale presente nel contesto dell'abitato.

e quello residuale delle piccole realtà, in particolare di quelle montane, nelle quali anche dal punto di vista culturale, oltre che per il pregio ambientale e naturalistico, va tutelata e incentivata la fruizione dell'ambiente naturale, così come si è perpetuato negli anni e così come è stato conservato dalle popolazioni. Si tratta di un intervento per la

clima di concordia e di condivisione sui contenuti della normativa, che giunge quindi in Aula in un quadro di elevato e allargato consenso.

la sua ragionevolezza, sapendo che su questo tema - condivido gli interventi dei colleghi - non possiamo permetterci una serie di normative-manifesto, ma dobbiamo garantire principi corretti e giusti

«La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, alle seguenti condizioni: all'articolo 4, i compiti assegnati a Regioni, Province e Comuni per lo sviluppo degli spazi verdi urbani siano formulati come facoltà, attenuando così il carattere impositivo delle disposizioni ivi previste, al fine di tutelare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali; all'articolo 5, le competenze a carico delle amministrazioni comunali ivi previste siano formulate come facoltà e non come obblighi, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali. Si segnala, inoltre, all'articolo 1, comma 2, l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni sia nella realizzazione delle iniziative di promozione per la conoscenza dell'ecosistema boschivo, sia nella definizione della modalità di realizzazione della messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone. Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza,

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione che sull'articolo 6, sul quale il parere è di semplice contrarietà».

2.101, 3.101 e 6.0.100, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime poi parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.102».

parere conforme al relatore

vengono inserite alla fine del comma 1 dell'articolo 1. Quindi, si accoglie l'emendamento con questa riformulazione che viene collocata alla fine del comma 1 dell'articolo 1.

che la messa a dimora di un albero possa essere dedicata anche a minori adottati.

grazie al Gruppo del Partito Democratico in Commissione. Tutto questo va bene ma, ai fini del perseguimento degli obiettivi generali, non possono e non devono essere trascurati il censimento, il rispetto e l'adeguata gestione degli alberi esistenti. Nella pratica corrente si osserva sovente come i Comuni si applichino talvolta per effettuare nuove piantumazioni ma, allo stesso tempo, ignorino il patrimonio verde esistente, ovvero devastino le alberature esistenti, molto più funzionali rispetto ai servizi ecosistemici esplicati,

La crisi della biodiversità è una delle principali emergenze del nostro pianeta e naturalmente interessa anche il nostro Paese, che pure è stato a lungo il secondo in Europa per il suo patrimonio di vita animale. Numerosi e noti sono i fattori che la determinano: deforestazione, distruzione degli *habitat*, inquinamento, agricoltura intensiva e quant'altro, e oggi anche l'Italia registra un calo preoccupante delle popolazioni naturali, in particolare dell'avifauna.

L'avanzata di asfalto e cemento, che ogni anno cancella boschi e campagne, è una realtà incontrovertibile. Mancano ancora gli strumenti legislativi che hanno portato altri Paesi europei all'adozione di politiche capaci di salvare il territorio e le sue risorse naturali. In questo contesto, con una progressiva urbanizzazione, anzi uno sviluppo sempre più forte dei sistemi urbani, occorre curare in modo particolare la capacità di accoglienza che le nostre città debbono rivolgere alle altre specie. Ciò può essere fatto attraverso una politica verde che sappia, tra l'altro, tutelare e arricchire il patrimonio vegetale (alberi, alberate, siepi), con interventi edilizi che permettano ancora la nidificazione di tanti animali senza quella uniformità di costruzioni che negano cavità, anfratti e aperture in cui sia possibile la riproduzione degli uccelli. Il sistema arboreo è fondamentale: ogni albero rappresenta una fonte di vita, per quanto riguarda non solo la riproduzione ma anche le risorse alimentari, e questo ci dovrebbe sollecitare a curare in modo particolare il nostro patrimonio di alberi. Tra le azioni positive che possiamo condurre con semplicità c'è indubbiamente l'individuazione dei tempi opportuni per eventuali operazioni di potature e, se necessario, di tagli e abbattimenti. Questi devono essere condotti nei periodi di riposo della vegetazione e al di fuori delle fasi biologicamente più importanti e delicate

Anche l'Europa con due direttive - la direttiva 79/409 CEE (uccelli) e la direttiva 43/85 (*habitat*) - ha richiamato gli Stati membri alla necessità di conservazione e tutela degli animali selvatici, soprattutto durante la nidificazione, la riproduzione e la dipendenza dei piccoli nati dai genitori. La legge n. 157 del 1992 ha vietato inoltre ogni forma di danneggiamento e distruzione dei nidi, delle uova e dei piccoli. Dunque, eventi traumatici come le potature o gli abbattimenti non possono essere condotti in primavera e in parte dell'estate, dal momento che diverse specie hanno anche una seconda nidificazione. Non può sfuggire come non sia solo il fare a pezzi un albero capace di distruggere la possibilità di perpetuare la riproduzione; spesso i nidi sono abbandonati durante la cova anche a causa del disturbo biologico, vale a dire del rumore e della "aggressione" che subiscono gli alberi anche vicini a quello in cui è in corso la nidificazione. Questo emendamento raccoglie dunque il dettato delle direttive europee e della legge nazionale ed è teso anche ad evitare i contenziosi aspri che spesso si verificano tra cittadini associazioni, da una parte, ed amministratori indifferenti o distratti dall'altra. La Convenzione di Rio sulla biodiversità diviene realtà proprio se siamo capaci di adottare comportamenti quotidiani, anche piccoli, che rendano possibile la convivenza tra la nostra specie e le altre, con l'esercizio di un sereno senso di responsabilità.

e vissuti i parchi e gli spazi verdi all'interno delle nostre città. Chi, infatti, più dei bambini che frequentano i parchi e gli spazi-giochi attrezzati,

Si richiede che essi vengano tutelati quali strumenti fondamentali per la conservazione della biodiversità, ai sensi delle diverse direttive europee direttive uccelli e *habitat,* già citate, in parte modificate e poi recepite con le leggi italiane). Anche gli spazi verdi urbani sono in realtà, in alcuni casi, delle reti ecologiche e dei corridoi biologici. Roma ne un esempio con i grandi parchi che esistono. Anche la Conferenza di Nagoya, tenutasi nell'autunno scorso in Giappone, ha voluto richiamare i Paesi della terra a far fronte alla crisi della biodiversità che, a causa degli interventi dell'uomo sulla realtà che lo circonda, cancellano ogni giorno *habitat* e la stessa possibilità di vita per tante specie. Si prevede che nei prossimi anni si rischi di perdere un quarto dei mammiferi e un terzo dell'avifauna del pianeta. Questo bollettino di quella che potremmo definire una guerra alla natura, di cui non siamo tutti a volte pienamente consapevoli, richiede delle risposte responsabili e concrete, anche nel nostro Paese. Ho già avuto modo di accennare alla perdita di biodiversità che l'Italia subisce - una morte quotidiana e silenziosa, gravissima - dovuta in modo particolare alla cancellazione di ecosistemi, che invece politiche più accorte ed obbedienti alle direttive internazionali potrebbero evitare. Una politica intelligente e praticabile è senza dubbio quella della tutela delle reti ecologiche e dei corridoi biologici, vale a dire di quel sistema di aree ancora verdi, ricche di biodiversità animale e vegetale, che sopravvivono nelle nostre città e che devono essere collegate tra di loro per permettere lo spostamento degli animali, il loro incontro e la loro in poche parole, la sopravvivenza di tante forme di vita. Infatti, alla connessione (cioè alla messa in rete) si oppone la frammentazione che porta all'estinzione delle popolazioni locali, prigioniere dei loro sempre più ristretti territori. La funzione delle reti ecologiche e dei corridoi biologici che le pongono in connessione è uno strumento primario che ogni forma di urbanizzazione dovrebbe rispettare ed anzi tutelare; senza voler qui sottolineare come la nostra stessa qualità della vita, la vivibilità delle nostre città e il diritto alla salute passino attraverso le stesse misure che consentono la sopravvivenza alle altre specie. Quello all'ambiente è ormai in letteratura giuridica riconosciuto come diritto diffuso ed ha una valenza sociale enorme, come sanno bene i cittadini che nei sistemi urbani più soffocati da asfalto e cemento pagano prezzi altissimi all'inquinamento, al rumore, alle isole di calore e alla mancanza di verde. Ritengo che l'emendamento 3.102 (testo corretto) sia perfettamente rispondente allo spirito del provvedimento che, partendo dal disegno di legge del Governo, è stato opportunamente dotato dalla Commissione ambiente di un più ampio e sacrosanto respiro. Le modifiche apportate rivelano, infatti, un'esigenza di inquadrare in modo più vasto le realtà urbane, e penso che l'approvazione della tutela delle reti ecologiche e dei corridoi biologici sia una misura necessaria e coerente a questo progetto.

volto a prevedere che le disposizioni della legge vengano estese ad arbusti, cespugli e siepi di interesse ecologico e naturalistico presenti nell'area urbana. L'importanza del verde urbano riguarda tanto il contributo che le aree verdi danno, e possono dare, in termini di fruizione del verde da parte dei cittadini e, dunque, di vivibilità della città, ma anche il contributo in termini ambientali, ecologici e naturalistici. occorrerebbe un riconoscimento e una maggiore consapevolezza generale di come il verde urbano si inserisce nel contesto dell'ecosistema urbano e delle relazioni esistenti con la fauna, ai fini dell'incremento e della valorizzazione della biodiversità urbana. In questo senso, un ruolo fondamentale è certamente svolto Tuttavia, grande rilevanza è ricoperta anche dagli altri elementi verdi, quali cespugli, siepi ed arbusti, che spesso detengono un alto valore naturalistico. L'emendamento 6.0.100 intende, quindi, includere nelle previsioni della legge questi altri elementi verdi, ovvero gli arbusti, i cespugli e le siepi presenti nell'area urbana e che abbiano un interesse ecologico e naturalistico. Avrete letto nei giorni scorsi articoli e «speciali» su come stiano scomparendo le farfalle.

esigente - e sulla tipologia dell'albero che viene messo a dimora. La seconda parte dell'emendamento credo sia utile. Non fa capo a nessun tipo di spesa da parte delle amministrazioni pubbliche

o commemorative. Nelle culture di molti Paesi si conoscono avvenimenti di questo tipo che rappresentano, soprattutto in piccole comunità o quartieri, momenti significativi di rapporto delle persone con la natura e anche di celebrazione o memoria o memoria di personalità significative per la comunità. Si tratta di un legame antico che si può rinnovare e che il Comune stabilisce attraverso una procedura di messa a dimora di alberi, quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri sono posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative.

ma poi trascurato dalle amministrazioni locali, cioè quello della piantumazione di un albero per ogni bambino nato

intervengo solo per sottolineare ed evidenziare il voto favorevole del Gruppo di Coesione Nazionale, con qualche punta di scetticismo in più rispetto al rischio

evidente che il richiamo ad una facoltà, per quanto legittimato dal riferimento all'autonomia dei Comuni, rischia di rendere la normativa meno impegnativa e di farle perdere una delle caratterizzazioni fondamentali. In conclusione, signor Presidente, che il confronto animato da questo provvedimento debba trovare ulteriore approfondimento rispetto al tema più generale della

trasformando la spesa corrente in spesa in conto capitale, e quindi collocandosi nel dibattito magari in materia di federalismo municipale, si corre il rischio di non determinare l'operatività reale delle norme che il Parlamento produce positivamente, come nel caso di specie.

Grazie Signor Presidente, come si può non condividere le disposizioni contenute in questo disegno di legge? Migliorare la qualità della vita nelle nostre città attraverso l'incremento del verde vuol dire salvaguardare la nostra salute e quella dell'intero pianeta e concorrere a cambiare in meglio lo scenario urbano che ci circonda, troppo spesso violentato

Il verde quindi come polmone, il verde come strumento per rendere migliore la qualità dell'aria: un singolo albero è in grado di fornire abbastanza ossigeno per dieci persone e di assorbire, a seconda delle dimensioni,

Inoltre, in una Nazione come la nostra, interessata per la maggior parte da fragilità idrogeologica, come purtroppo ci testimoniano le cronache delle ormai ordinarie tragedie dovute a frane ed esondazioni, spesso causate dalla mano dell'uomo che aggredisce il territorio attraverso un feroce disboscamento, promuovere il rispetto del patrimonio naturale e incentivare l'attività di piantumazione è un valido strumento di prevenzione del dissesto idrogeologico. L'Italia si scopre sempre fragile: troppo cemento lungo i corsi d'acqua così come a ridosso di versanti franosi, mentre ancora è grave il ritardo nelle attività di prevenzione. Sono ben 6.633 i Comuni italiani in cui sono presenti aree ad alta criticità idrogeologica: una fragilità endemica che non risparmia nessuna Regione italiana. Dati confortanti - è bene ricordarlo - arrivano invece dalle attività svolte nell'organizzazione del sistema locale di protezione civile. In tal senso, l'obbligo, già previsto dalla legge n. 113 del 1992, in capo ai Comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di ogni neonato residente, dovrebbe tradursi in una valida azione che concorra alla previsione e prevenzione del rischio idrogeologico. necessariamente inserirsi in una strategia più ampia; ovvero, per ovviare ai rischi sopra descritti è necessario innanzitutto promuovere una cultura ambientalista attraverso la divulgazione della conoscenza dei temi della sostenibilità ambientale e la diffusione delle azioni volte ad arricchire il patrimonio naturale. Essenziale risulta a tal fine il coinvolgimento delle giovani generazioni affinché si orientino verso scelte sostenibili. In questo senso si colloca il recupero e il rinvigorimento della tradizione di festeggiare la «Festa degli alberi» attraverso l'istituzione della «Giornata nazionale degli alberi» al fine di valorizzare l'ambiente e il patrimonio arboreo e boschivo. Il sistema economico poi non dovrebbe essere esente da questo impegno di tutela ambientale: ben vengano, quindi, misure che promuovano la sinergia fra pubblico e privato contenute nel disegno di legge, specie nelle aree urbane, attraverso contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione al fine di promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo. La possibilità poi contenuta nel disegno di legge di detrarre le spese sostenute per il verde pubblico non può che rappresentare un valido incoraggiamento. Il testo è frutto di una serie di modifiche ed integrazioni, che sono risultate opportune al termine di un confronto diligente ed approfondito, che ha visto i Gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione,

i romani avevano istituito la giornata della messa a dimora degli alberi, una festa denominata *Lucaria*; alla fine dell'Ottocento, i nascenti Stati Uniti d'America, a partire da uno Stato pieno di boschi, il Nebraska, avevano istituito l'«*Arbor Day*», la giornata dell'albero; fu per primo Guido Baccelli, Ministro della pubblica istruzione, alla fine dell'Ottocento, a creare una Festa dell'albero, e poi fu Mussolini

di coinvolgimento nelle scuole, tra le giovani generazioni e nelle amministrazioni civiche. La seconda parte del disegno di legge aggiorna la legge n. 113 del 1992,

dell'amministrazione, in modo che alla fine del mandato di un sindaco si dica di quanto si è accresciuto il patrimonio arboreo nella sua comunità, permette di instaurare una verifica. È un atto tutt'altro che marginale. Voglio sottolineare che una delle modifiche che l'Assemblea ha accolto permette di aggiungere all'attività dei Comuni, che in molti casi sono limitate per le disponibilità economiche, attività di privati, di associazioni, di gruppi di cittadini che vogliano dedicare degli alberi e la loro messa a dimora, in particolare in contesti urbani, per finalità celebrative o commemorative. Dunque, si tratta di una iniziativa significativa. Se la legge n. 113 fosse stata applicata interamente, forse oggi avremmo in Italia 7 milioni di alberi in più. Tuttavia, ne sono stati messi a dimora diversi milioni, e penso che, se questa legge consentirà sia di celebrare una giornata degli alberi con forte partecipazione formativa per la cultura ambientale e per l'amore verso la nostra comunità, sia

che ha una valenza simbolica e certamente è molto positivo.

Presidente, colleghi, come relatore, ho approfondito anche le tematiche del mondo "verde" e dico subito che il Gruppo della Lega Nord che mi onoro di rappresentare voterà a favore di questo provvedimento.

alberi che il mio Comune attuava con le scuole elementari mettendoli a dimora, ma mi è capitato anche di vedere degli alberi famosi che avevano smesso la loro vita.

finestra"). Colleghi, vi invito di nuovo a cercare di non superare con il brusìo le dichiarazioni di voto. È un problema di decoro dell'Aula che riguarda la maggioranza e le opposizioni.

Grazie apparentemente non ha bisogno di molte spiegazioni: essi hanno una grande importanza dal punto di vista ambientale perché trattengono l'inquinamento, perché assorbono anidride carbonica, perché nelle città sono l'arma più efficace contro le isole di calore, cioè contro il differenziale termico che rende tutti i centri urbani più caldi di 1, 2, 3 gradi rispetto alle campagne circostanti. Ma il valore degli alberi (e questo credo che sia correttamente e con merito rilevato nel disegno

Intanto, perché le città con più verde urbano sono più vivibili, più sicure, con più spazi comuni per la vita collettiva. Così, non è un caso che i gruppi, i comitati, le associazioni che si battono contro il degrado di tante nostre periferie chiedano spesso, tra le risposte più urgenti, proprio la realizzazione di un nuovo parco cittadino, la risistemazione di uno spazio verde abbandonato e magari chiuso all'uso pubblico. Da questo punto di vista, la situazione dell'Italia è molto contraddittoria: ci sono nel nostro Paese città dove la dotazione *pro capite* di verde urbano è collocata sui migliori standard europei, ma ci sono anche quasi trenta Comuni capoluogo - cioè poco meno di un terzo del totale dei Comuni capoluogo - dove il verde urbano per abitante è sotto i cinque metri quadrati, dunque ben lontano da quanto prevedono gli standard urbanistici nazionali. Infine, in Italia più che mai, gli alberi di città tra hanno un valore culturale di straordinario rilievo. In alcuni casi, gli alberi hanno persino un alto valore morale, come nel caso dei Giardini dei Giusti sorti a Gerusalemme, e poi in molte altre città del mondo, per ricordare, collegandone la memoria ad ogni nuovo albero, donne e uomini che hanno speso la loro vita al servizio dell'umanità. Il nostro, signor Presidente, colleghi, è da sempre un Paese a vocazione urbana, nel quale il paesaggio è fatto di un intreccio, molto difficile da Gli alberi di città sono uno dei simboli più efficaci di questa doppia valenza, naturale e culturale, del paesaggio italiano, e spesso ne incarnano, altrettanto bene dei monumenti, delle piazze, dei palazzi storici, l'identità. Basta del resto citare del resto citare qualche esempio, conosciuto, credo, da gran parte degli italiani: dalla Quercia del Tasso sul Gianicolo a Roma all'Orto botanico di Palermo, con i suoi *ficus* di oltre 20 metri di circonferenza; dalla Pineta di Ravenna, che fu oggetto più di un secolo fa di quella che è stata forse la prima legge italiana di tutela ambientale, alle ville storiche della città di Roma, strappate faticosamente al cemento negli anni del *boom* edilizio. Proprio questa considerazione ha spinto il nostro Gruppo a proporre in Commissione ambiente una integrazione al disegno di legge che discutiamo, che è stata accolta e che per noi riveste un grande rilievo. Mi riferisco all'articolo 6, che introduce per la prima volta in Italia una tutela generale per gli alberi monumentali, cioè per quegli alberi da salvaguardare per la loro maestosità e longevità, per la loro rarità botanica o il loro pregio naturalistico, ma anche perché rimandano a eventi o a memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali. Molti di noi, credo, hanno in mente esempi più o meno corposi nei quali questo o quell'intervento edilizio o di risistemazione urbana ha comportato il sacrificio di alberi così. Questa norma, senza toccare le competenze di Regioni e Comuni in materia di gestione urbanistica, consente per la prima volta - di cominciare a mettere in cassaforte un patrimonio prezioso e spesso irriproducibile. L'articolo 6 è una delle ragioni, non l'unica ma una delle principali, per cui il Gruppo del Partito Democratico sostiene questo disegno di legge, e con convinzione voterà

ritengo importante informare la Presidenza e l'Assemblea del seguito dell'iniziativa dei molti senatori che hanno tentato la settimana scorsa di recarsi, per svolgere funzioni di sindacato ispettivo, nei centri di accoglienza immigrati nel Sud del nostro Paese. Nessuno di noi la settimana scorsa ha avuto accesso In seguito a quelle nostre iniziative, e anche all'interessamento della Presidenza, mi è stato possibile visitare ieri il centro di accoglienza di Santa Maria Capua Vetere, in Campania, dove sono di fatto detenuti 1.000 giovani tunisini.

che sono stata l'unica parlamentare a poter entrare ieri all'interno di questo campo. Ora, all'interno di una struttura che già di per sé è un carcere militare, c'è una doppia recinzione di rete metallica, e 1.000 giovani vengono tenuti sotto le tende per l'intera giornata. A 200 di loro il ministro Maroni ha promesso, qui nella nostra

di quello che era evidentemente un minore; la Polizia, molto zelante, mi ha risposto: «Ha tentato di fregare anche noi, senatrice, ma ha 18 anni e quindi resta qui». Era un ragazzo chiaramente spaurito, giovanissimo, che poteva benissimo essere indirizzato ai servizi del territorio. a conoscenza di tre casi: un ragazzo sposato, con tanto di certificato di matrimonio, con una giovane cittadina napoletana, che aspettava di unirsi a lui, e che non veniva rilasciato; un ragazzo sposato con una giovane tunisina, residente a Modena, e che non veniva rilasciato;

La notte precedente un gruppo di giovani ha tentato di evadere: si sono rotti gambe e quant'altro (infatti molti erano ingessati) e sono stati riportati nel campo. Mi chiedo

Perché non è possibile porre in essere altri procedimenti per l'identificazione, e abbiamo bisogno di creare questi autentici *lager*? perché non creare dei tavoli di partenariato, come si è fatto in occasione del Kosovo, e, visto che queste persone avranno il permesso di soggiorno, porre

La ringrazio, senatrice Carloni, per questa sua visita e per questa sua testimonianza, che rimane all'attenzione dei senatori presenti

Ha fatto bene ieri l'assessore Russo a chiedere la revoca incondizionata dei pedaggi autostradali, convocando i sindaci dei Comuni siciliani. La rete stradale siciliana non è pronta a sostituire il ruolo, anche se limitato, delle autostrade, perché quelle non sono ancora autostrade: ma si può immaginare un casello per il pedaggio alla fine della circonvallazione a Palermo, a Catania o a Trapani? Le file di auto condizionerebbero tutti i flussi di traffico delle grandi città e si recherebbe un danno a tutta la Sicilia.

Il pedaggio condizionerebbe i costi del trasporto delle merci in una Regione che vive, più di altre, una crisi economica ed occupazionale mai registrata prima. Per questo motivo intendiamo avvalerci anche dello strumento del sindacato ispettivo, per fare in modo che quanto meno

tutta la mia approvazione per quanto riguarda il rispetto della natura, l'arredo urbano, gli alberi e la festa degli alberi; tuttavia, di fronte a ciò che sta accadendo

nostro Parlamento non ha altro da fare che continuare ad occuparsi di mozioni che vengono rispolverate all'ultimo momento? Peraltro, non si occupa di mozioni anche recenti e di drammatica urgenza,

che il Presidente del Consiglio ed il Ministro degli affari esteri venissero a relazionare in quest'Aula sulla nostra politica estera, sul rapporto con l'Unione europea, sullo schiaffo sonoro che l'Italia ha preso a Lussemburgo, sulla mancanza di solidarietà dei Paesi del Nord Europa nei confronti del problema italiano degli immigrati,

per questa delicata fase della politica internazionale che sta vivendo il nostro Paese, oltre che a livello nazionale.

*(IdV)*. Signor Presidente, sollecito risposte ad interrogazioni che riguardano il sistema di riscossione da parte di Equitalia, Gerit ed altre società

Migliaia di cittadini scoprono che Equitalia, Gerit ed altre società iscrivono ipoteche sulle loro abitazioni per somme inferiori a quelle previste dalla legge. Ci sono ultraottantenni che hanno sempre adempiuto al loro obbligo fiscale, i quali improvvisamente scoprono di avere i loro beni immobili ipotecati e devono iniziare un calvario per ottenere giustizia. Voglio ricordare anche ai colleghi - molti si stupiscono perché non intervengo sulle banche - che la Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 4077 del 16 febbraio 2010, ha sancito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per un importo inferiore a 8.000 euro. Il fondamento giuridico della scelta compiuta dalla Corte suprema è che l'iscrizione di ipoteca è un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare e, in quanto tale, ne eredita le regole. Questo orientamento dichiara di fatto illegittimi e nulli milioni di procedimenti d'ipoteca esattoriale, ossia tutte le ipoteche finora iscritte a danno dei contribuenti e restituisce giustizia ai cittadini. Richiedere tributi prescritti, inviare cartelle esattoriali non dovute e iscrivere ipoteche per importi inferiori a 8.000 euro nonostante quanto ha affermato la Corte, oltre a mettere in moto un meccanismo perverso in aperta violazione dello statuto dei diritti del contribuente, impone al cittadino l'inizio di una vera e propria *via crucis*, con perdite di intere giornate lavorative, configurando il reato di estorsione quando per piccoli importi il contribuente si vede addirittura costretto a pagare due volte, piuttosto che iniziare l'onerosa pratica fatta di code interminabili presso gli uffici di Equitalia, Gerit e altre società per poter effettuare la contestazione. Ringrazio dell'attenzione

la cancellazione dei fermi illegittimi, una maggiore trasparenza nelle richieste di pagamento (solleciti, diffide, intimazioni, avvisi, cartelle) e la cancellazione di cartelle basate su crediti già pagati, prescritti, annullati e inesistenti sono un atto di civiltà giuridica. Signor Presidente, la ringrazio e mi auguro che il Governo

Comunque, con una serie di direttive dei vari Ministeri competenti, negli anni è stata ampliata anche a questi luoghi per i parlamentari la prerogativa dell'indagine ispettiva, però è stata bloccata il 2 aprile scorso con una circolare del Ministero dell'interno. Grazie all'intervento svolto pubblicamente in Aula la settimana scorsa e alle insistenze di alcuni di noi, oggi si apprende che almeno in Campania è concesso l'ingresso

con telefonate registrate dalla RAI in diretta, davanti al CIE di Ponte Galeria la settimana scorsa), ma mi ha invitato a presentare un'interrogazione parlamentare. Ora, però, con gli sviluppi campani vi è un'ulteriore incertezza del diritto.

che interessa tante persone, molte di più rispetto ai parlamentari ma molte di meno rispetto agli italiani, che vivono nell'incertezza. Mi riferisco ai tunisini ai quali dovrebbe essere dato presto un permesso di soggiorno temporaneo. Concludo dicendo il perché di tutto questo, cioè che non si è compreso bene

che condivido in parte. Infatti, credo si debba specificare, o evidenziare, una parte delicata del problema. Ritengo non vi siano dubbi sull'esistenza del potere-dovere di ogni parlamentare di esercitare la sua facoltà (ripeto: potere-dovere) ispettiva,

alle carceri, anche di alta sicurezza, agli ospedali, alle scuole, alle università, evidentemente attraverso un comportamento corretto, chiedendo o avvisando il titolare responsabile dell'istituto. Mi sono recato a Manduria, come altri colleghi si sono recati nei luoghi dove sono sorti questi centri, e dal punto di vista della correttezza istituzionale ho avvisato e ho preso contatti con il prefetto, il quale, con immenso con immenso imbarazzo, mi ha comunicato di una direttiva del Ministro che vieterebbe l'accesso a chiunque, compresi i parlamentari. Parlo naturalmente a tutto il Senato, teoricamente, ma mi rivolgo alla Presidenza (perciò ho preso la parola): la Presidenza del Senato ci deve dire qualcosa in merito. Io ho presentato un'interrogazione insieme ad altri colleghi all'inizio della scorsa settimana, subito dopo i fatti di Manduria. che mi sono poi recato nel centro di Manduria dicendo al prefetto di riferire al Ministro che io ritenevo illegittimo il provvedimento emanato e, sulla base della illegittimità, con la forza della legge, sono andato al campo di Manduria, dove, ahimè, non solo non ho trovato nessuno che mi dicesse che non potevo accedere, ma ho trovato le porte aperte e una fuga generalizzata di 1.500 persone che erano andate via andate via disperdendosi nelle campagne, con tutti i potenziali pericoli che quest'azione sconsiderata da parte di chi aveva la responsabilità avrebbe potuto determinare. Ma questo è un altro aspetto della vicenda, pure compreso nella nostra interrogazione. A me sta a cuore che la Presidenza del Senato dica come la pensa. Io non aspetto la risposta del ministro Maroni, perché sono certo che, secondo le abitudini di questo Governo e di questi Ministri, noi rischiamo di avere una risposta, se la avremo, tra mesi. A me interessa sapere come la pensa il Presidente del Senato, di cui sono componente: se ritenga che la prerogativa del parlamentare possa

ritengo che possa costituire un abuso, signor Presidente, perché non ci sono state date le benché minime motivazioni sull'interruzione di questo che io chiamo l'esercizio di un potere-dovere ispettivo. La prova che mancasse la giustificazione sta in quanto le ho riferito a proposito di Manduria: che non solo non c'era nulla a vietare eventualmente il mio accesso, ma non c'era nessuno che controllasse gli ingressi di chiunque e le fughe di 1.500 persone. Credo che questo problema sia urgente e attendiamo da parte della Presidenza del Senato una risposta in merito.

da parte del Ministro dell'interno, un elemento di conoscenza più precisa della circolare, delle sue motivazioni e della sua gestione. Su quest'ultima questione, che è anche di natura politica, oltre che